22 ottobre non avranno luogo. Per il resto, rimane invariato il calendario già approvato: pertanto la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni, impegnate in particolare nell'esame dei documenti finanziari e del decreto-legge sugli obblighi comunitari. La discussione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio inizierà a partire dalla seduta pomeridiana di mercoledì 4 novembre, secondo i tempi già stabiliti.

Il 9 ottobre scorso un funzionario di Palazzo Chigi ha impedito ad un senatore della Repubblica di entrare nell'Ufficio stampa.

Sono state intercettate varie persone e, come risulta dalla Procura della Repubblica, anche l'onorevole Antonio Di Pietro.

A che titolo un senatore della Repubblica viene preso di peso e buttato fuori da Palazzo Chigi? A che titolo quella persona è lì? E chi la paga? parlando di un parlamentare, il senatore Pedica, che per Fondi ha condotto una battaglia straordinaria, con esiti negativi

dell'integrità del Parlamento e dell'integrità dei senatori. Preannunciamo, inoltre, di aver già depositato un'interrogazione al riguardo perché il Parlamento ha bisogno di essere tutelato in ognuno dei suoi membri, in tutti i suoi membri.

condanna a questo Governo che, non sciogliendo il Comune di Fondi per infiltrazioni mafiose, ha regalato la vittoria alla criminalità organizzata e a quei delinquenti

regalando alla criminalità organizzata la possibilità di operare, come ha fatto questa mattina con Fiore, si è aperto un precedente pericolosissimo, per il quale le associazioni mafiose si sentirebbero indirettamente autorizzate a delinquere

- è stato approvato dal ministro dell'interno Maroni, il quale per tanti e tanti mesi aveva affermato che quel Comune presentava evidenti infiltrazioni mafiose e non avrebbe mai pensato a farlo sciogliere se non per infiltrazioni mafiose, altrimenti

non potrà più essere rieletto, perché comunque ha già completato due mandati e dunque la magistratura farà il suo lavoro per quanto le compete. Questo è un Governo che della lotta alla mafia ha fatto anche una ragione di esistenza, visto che in un anno e mezzo di attività, sia nel pacchetto sicurezza, votato in quest'Aula a più riprese, fino al voto finale,

c'è stata una lotta senza quartiere anche nei confronti dei beni dei mafiosi, che sono stati colpiti come nessun Governo in passato ha fatto. Su questi temi dunque non accettiamo lezioni da nessuno, anche se non vogliamo alzare i toni nelle risposte: credo che un Governo come questo non abbia precedenti per la lotta alla mafia nella storia della nostra Repubblica.